colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

*(PdL)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, circa trent'anni fa fu approvata la legge n. 468 del 1978, che introdusse in Italia la sessione di bilancio,

determinato condizioni di scarso controllo e scarsa trasparenza dei conti pubblici. Chi, come me, ha partecipato a quel dibattito ricorda perfettamente le tre linee di analisi critica in quel momento, che pure fu considerato un passo positivo in avanti. La prima era relativa ai tempi non sincronizzati tra i documenti di programmazione economica e le decisioni da assumere: il DPEF fu collocato a giugno, in una situazione nella quale il quadro economico non era del tutto chiaro, come non era chiaro, perché non poteva esserlo, il conseguente quadro di finanza pubblica, per la sessione di bilancio che cominciava, invece, il 30 settembre, con la presentazione della legge finanziaria, e poi si prolungava per tutti i mesi successivi, sostanzialmente fino al Natale.

è l'aspetto che possiamo chiamare efficienza. Il secondo aspetto era quello della trasparenza: i documenti di di programmazione economica dovevano essere leggibili, quantomeno da parte del Parlamento (ed io aggiungo: anche da parte del comune cittadino che paga le tasse).

Ebbene, per non dilungarmi troppo, in quel momento la critica più forte che anche il sottoscritto esercitò, dall'esterno del Parlamento, ovviamente, fu il fatto che per il controllo della finanza pubblica si scelse esclusivamente il controllo dei saldi finanziari e non degli addendi: non, quindi, dell'entità della spesa e dell'entità delle entrate, ma soltanto i saldi finanziari. E anche allora, come oggi, si disse che era un passo in avanti, dopodiché i decreti di attuazione avrebbero corretto queste distorsioni. Signor Presidente, 31 anni fa purtroppo il deficit pubblico veleggiava attorno al 10 per cento del PIL, ma il debito pubblico era attorno al 60 per In questi trent'anni, non correggendo questi tre aspetti, guarda caso ci siamo ritrovati con un deficit pubblico che prima di entrare a Maastricht, prima della crisi del 1992-1993, ha continuato a veleggiare attorno all'8-10 per cento del prodotto interno lordo all'anno il debito pubblico, nel frattempo, è raddoppiato in rapporto al prodotto interno lordo, passando dal 60 al 120 recita l'articolo 81 della Costituzione. Questo è un mistero della Repubblica italiana: la Costituzione prevede che non ci possa essere nessuna spesa che non sia adeguatamente coperta, e noi ci ritroviamo con il raddoppio del debito pubblico; il che vuol dire una pesante ipoteca su tutte le future, oltre che la presente, generazione di italiani; il che vuol dire che ogni anno, il 1° gennaio, quest'Aula e la Camera discutono della finanza pubblica dovendo mettere da parte 100 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico. Questo è il modo con cui si procede. Abbiamo fatto - a mio parere - un ottimo lavoro nell'Aula del Senato; abbiamo lavorato tutti insieme. Non era un lavoro perfetto: a mio giudizio, il lavoro perfetto sarebbe stato quello di affidare ad un'autorità indipendente il controllo della finanza pubblica, la certificazione dei dati di bilancio;

questa legge di riforma non è un tecnicismo per quattro pazzi tecnici addetti ai lavori, ma è il cuore della democrazia, il cuore portante della politica, perché, se non si ha conoscenza dei dati, non si può avere scienza; si ha applicazione perversa della scienza per la manipolazione dei dati.

in quella sede, il primo aspetto, fortunatamente, è confermato. In altri termini, i tempi sono adeguati e i documenti di programmazione coincidono con i momenti della decisione. Questo primo punto portiamolo a casa. Però

che, insieme al senatore Maurizio Saia, ho presentato alcuni emendamenti puntuali, che non sono altro che il ripristino del testo votato nell'Aula del Senato.

pietra miliare di qualunque percorso di serietà e correttezza - aggiungo: di qualunque elemento di democrazia e di politica, e non di tecnicismi da ragionieri - è l'andamento tendenziale a legislazione vigente. Ebbene, dico qui in Aula ciò che il senatore Morando non ha detto ieri: i colleghi, e lei, signor Presidente, siamo tutti consapevoli di come vengono calcolati i numeri riferiti all'andamento tendenziale a legislazione vigente? Ve lo racconto: non è la previsione delle spese o delle entrate in base alle leggi, perché nel *computer* prima nelle carte e oggi nel *computer* - della Ragioneria generale dello Stato si introduce un *file* chiamato «coefficienti di realizzazione». praticamente vuol dire che se una legge prevede un spesa di 100, quella spesa non viene iscritta per 100, ma viene iscritta sulla base di una memoria storica che nessuno conosce, che solo gli uffici della Ragioneria conoscono e in base al pregresso si dice che dovrebbe essere 100, ma siccome è stato speso normalmente 30, il coefficiente di realizzazione è 30 e viene scritto 30.

non lo sa probabilmente neanche il Ministro dell'economia, meno che meno il Parlamento, e meno che meno i cittadini contribuenti. dato di riferimento non si chiariscono i criteri, la finanza pubblica è appesa per aria per chi ha la responsabilità delle decisioni di politica economica e dipende esclusivamente da chi ha la chiave del cassetto dentro La pressione fiscale è una scelta politica di fondo. L'opzione che avevamo adottato nell'Aula del Senato era quella di un'indicazione programmatica; nel testo della Camera si è introdotto «a fini conoscitivi», come se fosse una curiosità statistica. Infine, signor Presidente, è evidente che se, sia del tendenziale, sia del programmatico non si ha l'andamento separato delle entrate e delle spese pubbliche, ma soltanto il saldo, è del tutto inutile parlare di politica economica. Per esempio, se si parla di abbassare la pressione fiscale, è evidente che delle due l'una: o si aumenta il deficit pubblico o si taglia la spesa corrente. Ma se non conosco qual è il profilo della spesa e qual è il profilo delle entrate come faccio a parlare, eventualmente, Al collega Legnini rispondo questo: nell'ambito degli 800 miliardi di spesa pubblica, ben più dei 35 miliardi indicati sarebbero tagliabili.

dell'economia e della politica italiana e, spesso, aree grigie tra economia e politica. È una scelta politica, non una fattibilità tecnica quella del tagliare la spesa pubblica.

spesa corrente con entrate *una tantum,* né si sarebbe potuto ricorrere ad un debito verso i lavoratori chiamato TFR per coprire altre forme di spesa. Questi sono due esempi concreti

un tecnicismo da addetti ai lavori: è il cuore portante della democrazia, della politica, della chiarezza, trasparenza e certificazione della finanza pubblica, che rappresenta oltre la metà

è presente in tribuna, in occasione della loro visita al Senato, una delegazione di studenti del liceo classico statale «Platone» di Roma. A loro rivolgo gli auguri per le prossime feste e, soprattutto, per le loro attività di studio.

alla luce del dibattito svolto in quest'Aula, posso serenamente riconfermarle. In sostanza, credo che anche dopo il passaggio alla Camera dei deputati il disegno di legge non abbia perso le caratteristiche di fondo presenti nel testo licenziato in prima lettura al Senato.

in questo terzo passaggio, sulla base di due considerazioni di ordine politico. La prima è che, comunque, leggi di riforma come questa potrebbero,

che una legge di riforma così importante entri subito in vigore anche perché ci sono questioni che oggi sono determinate in via provvisoria penso per esempio a tutte le misure sul bilancio - che invece finalmente, con questo provvedimento, assumono nuovamente carattere legislativo. Qual è il significato importante di tutto ciò?

che naturalmente è uno dei punti fondamentali che caratterizzano questa legge di riforma. Ho già detto nella relazione che io stesso presenterò qualche ordine del giorno proprio nel senso di chiedere al Governo, nell'atto dell'applicazione di questa norma, se ci sono innovazioni che possono essere ancora introdotte sul piano concreto;

Al riguardo il senatore Massimo Garavaglia ha introdotto una possibile idea che va sperimentata concretamente, quella cioè che le Commissioni bilancio si occupino seriamente, a partire dall'anno prossimo, di questo problema, cioè delle metodologie di

i problemi posti possono trovare soluzione. Vale lo stesso per alcune questioni tecniche, quali quella delle spese non ricorrenti o altre che certamente potranno costituire occasione di una ulteriore

su ciò che gli viene sottoposto per la decisione e dei poteri di controllo per quanto riguarda non soltanto i criteri di elaborazione ma anche i metodi di appostazione e di scelta che il Governo fa con il bilancio.

ci sarà una legge di stabilità, in cui le grandezze macroeconomiche saranno assolutamente e tranquillamente evidenziate, ed un collegato per lo sviluppo che si configura come il necessario completamente di una manovra ben fatta. Questo mi pare sia l'impianto complessivo della legge.

sarà la sede espressione di tutti i livelli politici e istituzionali che vanno a comporre l'aggregato pubblica amministrazione e che, quindi, nel Senato federale vi sia un impianto di coordinamento dell'intera finanza pubblica, che poi troverà la sua specifica applicazione ai vari livelli politici ed istituzionali che l'attuale Costituzione prevede. Mi pare che questo un contributo serio che l'intero Senato ha dato a questa legge, la cui approvazione costituirà il miglior suggello del lavoro fatto,

sia condivisibile. Francamente sono rimasto stupito da queste affermazioni perché - come spesso accade - si è vista la trave senza invece rendersi conto che forse si tratta solo di una pagliuzza. È tutto male quello che ci viene dalla Camera? È proprio così?

Quindi, a mio sommesso avviso, sarebbe assolutamente poco comprensibile se il Senato mutasse quell'atteggiamento che aveva visto una concordia di tutti i Gruppi politici su un testo condiviso e condivisibile e che non è mutato, se non per qualche miglioramento apportato dall'altro ramo del Parlamento.

di una riforma di ampia portata, che contiene anche delle deleghe, per cui il Parlamento avrà modo di ragionarci nel tempo, ma è opportuno che entri in vigore il 1° gennaio dell'anno prossimo. È un testo che mette insieme i rapporti tra Parlamento e Governo come mai era stato nel passato e divide i compiti

alla legge di contabilità del 1923, adeguando i rapporti tra Parlamento e Governo, suddividendo i rispettivi compiti e facendo in modo che il principio di responsabilità, che non è mai stato applicato nel nostro Paese e che ha portato tanti guai - basti ricordare l'esplosione del debito a seguito delle commistioni di responsabilità che esistevano nella cosiddetta prima Repubblica - possa finalmente trovare applicazione. Quindi, credo che questo testo, che è migliorativo rispetto a quello approvato dal Senato, sia importante e costituisca una grande riforma di struttura che ha tanto più senso in quanto possa essere accolta da tutte le parti del Parlamento, perché si tratta di regole che presiedono al lavoro dell'intera comunità del Paese. È una riforma strutturale e una riforma coraggiosa,

più efficiente da parte dell'amministrazione. È, inoltre, una riforma rispettosa dei reciproci ruoli di Governo e Parlamento, nella consapevolezza che la responsabilità deve essere attribuita a un soggetto per evitare scarichi di responsabilità che hanno portato tanti danni nel passato. Certamente la riforma non è una condizione sufficiente per il risanamento dei conti pubblici, ma ne è la condizione necessaria: senza un saldo sistema di contabilità pubblica non è possibile risanare i conti del Paese. È quindi lo strumento indispensabile per ridare vigore ai conti, per mostrare ai mercati internazionali quali sono le vere volontà del nostro Paese e, quindi, per compiere una grande riforma di portata anche internazionale che dia un senso a ciò che stiamo facendo tutti insieme. E qui ringrazio non la parte governativa e la maggioranza, ma anche l'opposizione e l'intero Parlamento. È una riforma indispensabile, infine, per applicare il federalismo fiscale, che credo sia un passo fondamentale per la modernizzazione del Paese e anche per la considerazione del livello di spesa. Una domanda necessita di una risposta: le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono effettivamente dirompenti? Hanno denaturato la struttura del provvedimento? A mio avviso assolutamente no. Per quanto riguarda il tema principale - il tema dei temi - che è stato posto nel dibattito di ieri e di oggi, la trasparenza dei dati non ne risulta assolutamente minata.

citerò solo il caso della legge finanziaria per il 2008, quando la Ragioneria si oppose ad alcuni tentativi del Governo di introdurre norme non coperte, a dimostrazione del fatto che la Ragioneria è un organo neutro, come si suol dire, del Paese, e non è organo

un vantaggio per una maggiore funzionalità nei controlli, compito che finora è stato trascurato, ma che questa legge affida ad un Parlamento più efficiente rispetto al passato. Per quanto riguarda il così detto Servizio del bilancio, è evidente che, trattandosi di *interna corporis,* questo Servizio può essere meglio istituito con delibera parlamentare o con modifica del Regolamento piuttosto che con una legge. Tra l'altro, il Parlamento in questo modo garantirebbe la propria supremazia e la propria autonomia rispetto al Governo. Quindi, se si può fare con una modifica del Regolamento, perché il Parlamento non dovrebbe accettare la sfida di farlo, e meglio, rispetto a quanto sarebbe disposto con una legge?

dei difetti che si sono riscontrati nel passato. Insomma, questa è una sfida che il Parlamento si trova davanti e che saprà sicuramente vincere solo se non si abbandonerà a schematismi come quelli dei riferimenti normativi ad una legge che l'autorizza: questo, infatti, è un modo per perdere sovranità e non per guadagnarla.

È chiaro che la responsabilità governativa ha un senso: poco senso avrebbe delegare ad un soggetto esterno l'accertamento della bontà di quanto si fa. È un accertamento delegato esclusivamente al Governo al Governo e agli elettori. In caso contrario, andremmo nella direzione di un sistema sostanzialmente tecnocratico, che francamente ci porterebbe molto lontano dal sistema democratico che tutti, pur nell'imperfezione, andiamo perseguendo. Trasformeremmo, tra l'altro, il Governo, che è già soggetto al Patto di stabilità europeo, che già non ha la sovranità monetaria, che dipende dalla BCE, e che in questo caso perderebbe anche la sovranità sui conti pubblici, in null'altro che una buca delle lettere. Francamente per qualunque Governo, di qualunque Nazione, di qualunque colore politico, mi sembrerebbe un esito inaccettabile. Se permette, signor Presidente, vorrei rivolgermi direttamente al senatore Morando, con il quale, in questi anni, abbiamo condiviso, dalle diverse parti politiche, la necessità di rinnovare il nostro sistema di contabilità pubblica e con il quale da tempo abbiamo perseguito queste novità, tra l'altro lavorando anche insieme - non è assolutamente un segreto - alla redazione del testo al nostro esame e dei successivi emendamenti.

del Senato consente al Parlamento un intervento più incisivo rispetto a quello approvato dalla Camera: forse potrebbe rivedere la sua considerazione con un giudizio meno critico in assoluto, ma soprattutto meno critico tenendo conto del dato che, lei ha fatto riferimento ad una parte molto limitata, che non modifica la sostanza del problema, la sostanza del testo. Quest'ultimo - a mio sommesso avviso - esce dalla Camera dei deputati rafforzato e migliorato (anche il testo approvato

accaduto alla Camera, che dia il segno che il nostro Paese non è insensibile ai grandi problemi di struttura, ai problemi delle regole, soprattutto in un momento difficile come quello Non si giustificherebbe altrimenti - me lo lasci dire - una diversa presa di posizione rispetto a quanto è avvenuto alla Camera. Se fossero apportate delle modifiche, credo che la Camera dei deputati non starebbe inerte e non le recepirebbe molto facilmente. L'occasione odierna, in conclusione, signor Presidente, potrebbe forse servire anche per salutare la legge finanziaria che, nell'ultimo trentennio di travagliata vita repubblicana, croce e delizia dei conti pubblici, ci ha accompagnato. Essa con la nuova legge di stabilità finirà il suo *iter*, con la speranza che la legge di stabilità porti anche una considerazione migliore delle finanze pubbliche e costituisca lo strumento indispensabile per il loro risanamento, fine senza il quale fine senza il quale anche quella giustizia retributiva e redistributiva che molti inseguono non potrà essere conseguita. «La 1a Commissione permanente, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Presidente, se la parte dispositiva viene mantenuta integralmente possiamo accettare la proposta del Governo, anche sulla base di cosa a giudizio del Governo dovrebbe essere sfumato. Se, infatti, ad essere sfumate sono valutazioni che non incidono sul dispositivo finale, da parte nostra non ci sono problemi.

*(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.1 è teso a riproporre la costituzione della Commissione bicamerale per la trasparenza dei conti pubblici. Si tratta come ho cercato di spiegare ieri, sia pure senza grande capacità di convinzione nei confronti del Governo, come si è ascoltato questa mattina - di una questione di rilievo cruciale. Nel testo della Camera il senso della proposta del Senato viene stravolto per una ragione molto banale. Se si legge il testo dell'attuale articolo 4, così come ci viene dalla Camera dei deputati,

se si fosse trattato di controllo degli andamenti di finanza pubblica, certamente la proposta di costituire un'apposita Commissione bicamerale sarebbe stata da respingere, perché il controllo degli andamenti di finanza pubblica è, classicamente, una funzione specifica che, per quello che riguarda l'attività del Parlamento, viene svolta dalle Commissioni permanenti Sarebbe stato perciò assurdo proporre di espropriare e di spostare questa competenza dalle Commissioni permanenti ad una Commissione bicamerale da costituire *ad hoc*. Peccato, però, che nel testo del Senato non si parlasse mai di controllo degli andamenti di finanza pubblica, ma semplicemente della costituzione di una Commissione non per valutare atti del Governo in sede di gestione del bilancio, ma, al contrario, per occuparsi di una robusta iniezione di trasparenza

Sempre nel testo del Senato - e quindi anche nell'emendamento che noi qui riproponiamo - si fa riferimento all'introduzione di trasparenza nella elaborazione dei dati. E un punto è assolutamente cruciale: il testo della Camera, inesorabilmente, richiamandosi all'attività delle Commissioni bilancio permanenti, si riferisce sistematicamente ad atti del Governo, quelli previsti dall'articolo 3. Il testo del Senato non faceva minimamente riferimento ad alcun atto del Governo, proprio perché non si occupava di controllo degli andamenti di finanza pubblica, ma semplicemente di esaminare come i dati di finanza pubblica vengono elaborati, soprattutto in un'occasione. Colleghi, capisco che queste cose possono sembrare tecnicalità assurde, ma guardate che qui c'è la sostanza del rapporto tra Parlamento e Governo. La storia dei Parlamenti comincia decidendo su chi ha il potere di decidere sul bilancio. Il principio «nessuna tassazione senza rappresentanza» è il principio da cui nascono i Parlamenti. Attualmente, qual è il documento fondamentale nella nostra procedura di decisione di bilancio? È la redazione da parte del Governo del bilancio a legislazione vigente;

Non abbiamo perfetta cognizione di quali siano le metodologie di elaborazione e di raccolta dei dati,

È chiaro che noi non abbiamo cognizione delle metodologie di costruzione del dato del bilancio a legislazione vigente (voce per voce e nel complesso) e il risultato è che il documento base della decisione di bilancio non è dal Parlamento padroneggiabile sotto il profilo della sua attendibilità di partenza. Non è in questione la fiducia nel rapporto con il Governo *pro tempore*: è in questione la possibilità del Parlamento di decidere conoscendo. nasce l'esigenza di istituire la Commissione bicamerale sulla trasparenza: sulla trasparenza, non per il controllo degli andamenti di finanza pubblica. Avrebbe ragione da vendere la Camera se avesse abrogato una Commissione bicamerale volta a fare quello che devono fare e fanno abitualmente le Commissioni bilancio. La Commissione bicamerale che avevamo previsto e che riproponiamo con l'emendamento 4.1 esclusivamente rivolta ad accompagnare il processo di iniezione di trasparenza nella elaborazione e nella raccolta dei dati. Questo era l'unico obiettivo di questa Commissione, e per fare questo le Commissioni bilancio di Camera e Senato, così come sono, hanno limiti evidenti che risulteranno purtroppo - sarei contento di sbagliarmi - insormontabili. nasce la riproposizione della Commissione bicamerale. Signor Presidente, mi permetterà di esprimere un parere motivato su questa questione, che naturalmente è una delle più importanti perché la Camera, nel secondo passaggio, ha

il Governo ha svolto sul fatto che anche questa espunzione ha trovato alla Camera un'unanimità. Ciò di cui mi voglio occupare è di rispondere esattamente ai problemi posti dal senatore Morando.

effetti sicuramente migliori proprio nel rapporto tra Governo e Parlamento del quale mi sono occupato nella replica. Credo però che la soluzione data dalla Camera dei deputati non modifichi nel merito le norme

occuparsi esattamente dei problemi che sono stati posti. La seconda parte dell'osservazione del senatore Morando attiene alla

È un'obiezione che ha certamente un suo fondamento, perché le Commissioni bilancio naturalmente devono occuparsi anche di una serie di altre questioni.

può strutturarsi - ad esempio, con una sottocommissione *ad hoc* - per occuparsi di tale tema. È un esperimento che dobbiamo portare avanti a partire dal gennaio

di poter esercitare attività di controllo; non siamo nel campo dell'elaborazione di metodologie.

Chi la fa questa apposita intesa? In ogni caso, una volta approvata la legge, ci saranno grandi cervelloni che si metteranno a costruire l'apposita intesa. Passeranno mesi, passeranno anni, l'apposita intesa verrà prima ipotizzata e poi cambiata perché uno dei due contendenti non sarà d'accordo. Il risultato sarà che non vedremo mai più Ove mai, poi, alla fine tale collegamento venisse a stabilirsi, sarebbe ostacolato dalla seconda misura che la Camera ha introdotto, modificando una norma che prima diceva, in buona sostanza,

30 giorni dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* (cioè la cosa più normale), ma al giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti. Peccato che il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* lo conoscono tutti, il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Corte dei conti non lo conosce nessuno. Il risultato è che si ritarderà, con una scadenza che non si può controllare in modo trasparente. Queste modificazioni

- e lo dico seriamente - queste sono le classiche questioni, senatore Morando, sulle quali si potrà intervenire immediatamente nel caso in cui

parere del Governo

In questo momento in tutto il mondo la discussione di politica economica verte sul seguente problema:

molto espansive sotto il profilo monetario. È assolutamente assodato che questi interventi di tipo espansivo abbiano avuto il merito, sia dal lato delle politiche di bilancio, sia dal lato delle politiche monetarie, di ridurre la durata della crisi e facilitare l'avvio della ripresa. In questo momento, in tutto il mondo, i grandi esperti, gli uffici studi, i grandi istituti di ricerca si stanno misurando sul seguente problema: è del tutto evidente che occorre, che i Governi adottino politiche di progressiva restrizione di bilancio, perché non si può proseguire in una situazione nella quale i deficit pubblici sono esplosi come è accaduto nel corso dell'ultimo anno. In secondo la Banca centrale europea, la *Federal Reserve* e le altre grandi banche centrali rilevanti ai fini dell'andamento della politica monetaria di tipo globale stanno discutendo su quando cominciare a rendere più restrittiva la politica monetaria. Il nodo fondamentale da sciogliere è come si fa ad adottare queste due misure di rientro - solitamente si usa l'espressione *exit strategy*, anche in questo caso, per dire tornare indietro rispetto alle politiche espansive, sia dal lato monetario che da quello della politica di bilancio - senza uccidere il bambino, cioè senza fare precipitare di nuovo il mondo in una spirale recessiva. Si tratta di una questione anche teorica particolarmente difficile, che è stata affrontata nei giorni scorsi dal presidente Obama in un importante discorso alla Nazione sulla politica economica. Sapete qual é l'istituto di ricerca a cui ha fatto riferimento il presidente Obama per collocare la propria posizione e la propria valutazione su questo punto, che - ripeto - è oggi oggetto di confronto tra i massimi esperti di economia e i più grandi istituti di ricerca economica di tutto il mondo? É stato il *Congressional budget office*, il CBO americano, il Servizio del bilancio del Parlamento. Ciò che deve essere chiaro è che, a fronte di quella citazione, nessuno, né i repubblicani né i democratici, ha avuto da eccepire sul dato e sullo studio.

il suo carattere *bipartisan*, il suo "incistamento", il suo insediamento, nel Congresso americano, cioè nella sede del potere legislativo

in Italia abbiamo questo deficit. Non abbiamo una sede unificata del Parlamento che acquisisca progressivamente la stessa autorevolezza. Come ho cercato di dire ieri, questo deficit diventerà drammatico quando si tratterà di passare all'attuazione della legge sul federalismo, perché a quel punto - signor Presidente, sono disposto a fare scommesse! - litigheremo non sulle scelte politiche, ma sui dati, perché i dati saranno solo di parte governativa ed il Parlamento ed il sistema delle autonomie tenderanno a discutere della loro attendibilità.

e non ci siamo riusciti, ed il Vice Ministro sa che abbiamo provato, che abbiamo provato assieme e che abbiamo provato seriamente. Per cui l'appello lo rivolgo io a lei, signor Vice Ministro: cambi il parere su questo emendamento, almeno su questo creiamo una condizione di vincolo, altrimenti il Servizio del bilancio unificato non si farà, e lei sa bene che se non è previsto nella legge non si farà, e questo sarà un danno per la Nazione. Questa è la verità delle cose che nasce dall'esperienza. Non cambiate la legge su alcun altro aspetto se non volete cambiarla, anche se secondo me sarebbe ragionevole farlo, ma almeno su questo punto prendete una decisione che corrisponda all'orientamento unanime su questo punto eravamo stati unanimi in Commissione e in Aula, compreso il Gruppo dell'Italia dei Valori: avevamo tutti detto che ci voleva la struttura unificata. Possibile che questo Senato, che tre mesi fa ha detto all'unanimità che ci vuole la struttura unificata, adesso annoveri una larga maggioranza contraria a questa soluzione? Non accetto su questo punto l'accenno che ha fatto il vice ministro Vegas, e cioè che se anche solo su questo punto rimandiamo il testo alla Camera, la Camera non lo approverà più: questo atteggiamento non

*(PdL)*. Signor Presidente, approfitto per illustrare congiuntamente gli emendamenti 6.0.2, 10.4, 10.7

aggiuntivo. Signor Presidente, un carissimo amico, che ha calcato quest'Aula e quella della Camera e ha concluso la sua vita terrena cosciente nel seggio della Camera, 31 anni fa propose e promosse una discussione su questo argomento perfettamente sintetizzata ora dal senatore Morando. Si invitò a Roma il direttore generale del *Congressional Budget Office* americano per spiegare allora al Parlamento italiano quale fosse la funzione cruciale del Servizio di bilancio unificato. Mi dispiace, signor Presidente, ma il film che vedo oggi è un vecchio film di 31 anni fa: non mi è piaciuto allora

come lo è, se permette, signor Presidente, la non chiara coerenza di chi lo ha votato tre mesi fa e, magari, oggi è chiamato a non votarlo.

che vorrei sottoporre alla riflessione di quest'Aula e agli amici del PdL e della Lega: senza quella pietra miliare di chiarezza questa legge di conferma - e non di riforma - del bilancio dello Stato rischia di minare i fondamenti del federalismo fiscale, perché senza questi dati di riferimento voglio vedere quale tipo di dibattito potrà aprirsi, per esempio, sulla definizione dei costi standard. E se non vi è una definizione corretta dei costi standard, come applicheremo nel concreto quella grande riforma di responsabilità che si chiama federalismo fiscale? E non si dica che, dopo aver aspettato 30 anni, aspettare 30 anni e due mesi per fare una riforma vera è la fine del mondo, il diluvio universale! È vero, È vero, il Governo deve padroneggiare i dati di finanza pubblica, questo è fuori discussione. Il tema che mi permetto di sollevare e che altri colleghi hanno sollevato prima

che la Ragioneria negò al Governo Prodi e che il Governo Prodi tentò di aggirare con un lettera firmata dal sottosegretario Sartor. In quel momento prevalse (i colleghi ricorderanno certamente che condussi una battaglia in quel senso) l'opinione della Ragioneria, ma il tema è: questo bollino è autoreferente, è nell'incognita dei criteri con i quali, giustamente, la Ragioneria deve apporre i bollini, ma il Parlamento ed il Governo hanno il dovere, oltre che il diritto, di sapere quali sono i criteri previsti per l'applicazione del bollino della Ragioneria,

Sul piano della cassa è palesemente un aumento di fabbisogno di cassa, perché sono fondi non direttamente utilizzati che, se utilizzati per spese, diventano fabbisogno di cassa. Ma, sul piano della competenza, se quel debito è già assegnato a soggetti titolari del TFR, come fa a fornire una copertura di competenza ad altre voci di spesa? Questo è il tema, cari colleghi, non la responsabilità della Ragioneria dello Stato, qualunque sia il Governo, di certificare: il Parlamento ed il Governo debbono conoscere quali sono i criteri in base ai quali

La ringrazio, Presidente. Dicevo che, ove non si riesca a raggiungere in tempi rapidi l'intesa, anche all'interno di una sola Camera, qualche passo in avanti bisognerà farlo.

che la soluzione proposta dalla Camera lascia ancora margini e che l'attivazione di entrambe le Camere o addirittura di una sola può essere una strada percorribile,

di quei dati. Il mio parere pertanto è contrario, con l'auspicio che, come ho detto, già dal prossimo anno si cominci concretamente a trovare soluzione a questo problema. della burocrazia che sopravanza il Governo, allora il mio parere diventerebbe duramente contrario, perché potremmo dar luogo addirittura a due burocrazie che si scontrano tra di loro. Questo pericolo è evitato e ho una straordinaria fiducia nella capacità dei Governi di padroneggiare i dati

è violentemente contrario a questo testo e, ove esso venisse modificato, lo rimanderebbe indietro per una cosa che non ha nessuna ragione di esistere.

al pilastro su cui necessariamente si regge l'ambizione di un progetto di riforma della decisione di bilancio, adeguato ad un nuovo sistema istituzionale: quel sistema che si è andato profilando tra la prospettiva federalista, dentro un più esigente recinto europeo e, soprattutto, il configurarsi di un maggioritario ancora imperfetto, che è nato dal lato della riforma elettorale, ma che non ha ancora attuato conseguenti e coerenti adeguamenti del sistema Di questo stiamo parliamo. L'ambizione che esprime il progetto di riforma della contabilità, se manca il pilastro di un autorevole ed indipendente Servizio del bilancio parlamentare, manca dell'elemento essenziale

si discusse cioè della nascita del Servizio del bilancio. Sono stato sollecitato in questo da uno scritto del professor Marcello Degni, che allora faceva parte di quel gruppo di giovani

si capì che la riforma che introduceva la tipizzazione della legge finanziaria e la necessità della quantificazione degli oneri richiedeva un'apposita struttura parlamentare specializzata. Si discusse se dovesse essere questo un compito affidato alla Corte dei conti, ad un Servizio unico o ad un Servizio specifico per i due rami del Parlamento: si preferì lasciare la Corte dei conti fuori dal recinto delle decisioni parlamentari, ma le si affidò il referto di parificazione sui bilanci e si scelse la strada del Servizio «a due teste». Allora era una soluzione adeguata a quel momento storico ed istituzionale; ci si addentrava anche in un mondo inesplorato. Oggi invece l'esperienza che abbiamo alle spalle ci insegna, con evidenza palmare, che il motivo di tanti fallimenti nel controllo della finanza pubblica è la mancanza di una dialettica corretta tra Parlamento e Governo e nell'ambito di un ragionamento più ampio parliamo di riforme basate su uno scambio virtuoso tra Governo e Parlamento. I colleghi costituzionalisti mi scuseranno se uso una semplificazione, ma lo schema è questo: al Governo più poteri per governare in modo efficiente e per realizzare il proprio programma; al Parlamento più strumenti per esercitare in modo più penetrante la funzione di controllo. Lo ha ricordato per l'applicazione concreta al bilancio il presidente Azzollini: più spazio di decisione al Governo, ma, nella partita che resta di competenza del Parlamento, poteri e strumenti più penetranti. Lo strumento per realizzare questo scambio è esattamente la presenza di una struttura dotata di tutte le competenze tecniche, del peso scientifico e organizzativo, per interloquire alla pari con Governo e Ragioneria dello Stato. senatori Quagliariello, Zanda e agli altri colleghi che stanno lavorano alla modifica dei Regolamenti parlamentari, ancora una volta articolati sullo schema «poteri e tempi certi al Governo per la realizzazione del programma e garanzia all'opposizione di poter esercitare con strumenti adeguati il proprio ruolo di controllo»: ma a cosa state lavorando se per una delle funzioni più importanti del Parlamento, la sessione di bilancio, stiamo oggi decidendo che questa funzione non sarà quella che state prevedendo nelle proposte di modifica dei Regolamenti? Sarà dunque squilibrata, inadeguata, e quindi è inutile il lavoro che state facendo.

quella struttura dispone di 230 unità, non di qualche decina alla Camera e meno di una decina al Senato. Altro che *interna corporis*, vice ministro Vegas: è una scelta politica di fondo. Lì il 70 per cento dei funzionari sono economisti, c'è un *board* in cui le migliori menti economiche del Paese partecipano e danno il loro orientamento. Si dimostra che il sistema presidenziale resta interamente nell'ambito di un recinto di una democrazia vitale grazie a vigorosi contrappesi. Non vogliamo qui fare questo salto di qualità: si capisce che c'è un solo argomento per non farlo, che è quello della paura di toccare di toccare l'esistente, della pura conservazione dell'esistente, ma la conservazione dell'esistente dopo acclarati fallimenti non è mai una buona politica. Dite che si potrà fare egualmente? Vi attendiamo alla sfida. La promessa è stata già fatta qualche anno fa: il risultato è stato troppo modesto rispetto alle necessità di una buona conduzione della finanza pubblica e di una buona condizione - ha ragione il senatore Baldassarri di una democrazia parlamentare che non vuole impaludarsi in un gioco di veti reciproci tra Governo e Parlamento, tra maggioranza e opposizione, ma vuole dare fino in fondo il proprio contributo per il benessere del Paese.

comunico che nella giornata odierna è scomparso il dottor Giancarlo Morosetti, che per lunghi anni è stato uno stimato funzionario di Palazzo Madama e già direttore del Servizio di Segreteria e dell'Assemblea. pertanto alla sua famiglia e all'Amministrazione tutta del Senato i sentimenti del cordoglio e della vicinanza della Presidenza e di tutti i senatori. ora le decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, che si è riunita questa mattina ed ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 21 gennaio 2010. Per questa settimana resta confermato l'esame dei disegni di legge di contabilità e finanza pubblica, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, di conversione del decreto-legge sui concorsi per dirigenti scolastici, nonché le ratifiche di accordi internazionali, con l'integrazione delle mozioni sull'obesità infantile e sulla proliferazione delle armi nucleari. Per quanto riguarda la sessione di bilancio, non appena trasmessi dalla Camera dei deputati, i documenti finanziari saranno immediatamente assegnati alla 5a Commissione permanente e, in sede consultiva, alle altre Commissioni, che sono sin d'ora autorizzate a convocarsi fin dalla giornata di venerdì 18 dicembre. Le Commissioni dovranno trasmettere entro le ore 12 di lunedì 21 dicembre i propri rapporti alla Commissione bilancio, che riferirà alla Assemblea a partire dalle ore 18,30 dello stesso giorno. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 19 di lunedì 21 dicembre. L'esame dei documenti finanziari proseguirà in Assemblea nelle due sedute di martedì 22 dicembre, fino alla sua conclusione. Nella seduta pomeridiana di martedì 22 dicembre, si svolgerà la chiama per l'elezione di due senatori Segretari, a scrutinio segreto mediante schede. Successivamente le urne resteranno aperte. Dopo le votazioni finali, con la presenza del numero legale, dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, saranno discusse ratifiche di accordi internazionali definite in Commissione. L'Assemblea riprenderà i propri lavori alle ore 17 di martedì 12 gennaio 2010 con l'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi. Per la discussione del provvedimento i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi secondo un criterio che ha tenuto conto di reciproche esigenze e cessioni. Seguirà l'esame del disegno di legge sulle cure palliative, con eventuale seguito nella settimana successiva, a partire da martedì 19 gennaio. Nel corso di tale settimana il calendario prevede altresì la legge comunitaria per il 2009 e ulteriori ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione. Infine, il calendario del mese di gennaio potrà essere integrato con la relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia e con documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. **Programma dei lavori dell'Assemblea**

degli spazi di manovra in merito ad un annoso problema sul quale tutte le forze politiche e i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI si trovano d'accordo, ossia sulla necessità di un alleggerimento del Patto di stabilità.

nella sua stesura iniziale l'articolo 8 aveva previsto al comma 6, attraverso una piena condivisione fra maggioranza ed opposizione, ed opposizione, la possibilità che nell'ambito dei livelli massimi stabiliti per i vincoli del Patto di stabilità vi fosse la possibilità per le Regioni di adattare detti vincoli alle singole realtà comunali, municipali e provinciali, nonché di modulare anche la possibilità di una compensazione

gli effetti di vincolo sul Patto di stabilità. Si è quindi ottenuto un effetto *rebound* rispetto alla stesura iniziale, che prevedeva - e fu un articolo votato da tutto da tutto il Senato - un alleggerimento del Patto di stabilità interno; ora infatti, con l'abrogazione del comma 6 e il mantenimento invece del comma 4, si prevede che le spese in conto capitale la decisione di finanza pubblica stabilisce la quota di indebitamento articolata per Regioni e poi per singole amministrazioni locali. Ciò significa, di fatto, andare in una direzione opposta rispetto a quella verso la quale il Senato si era mosso in prima lettura. Il problema della necessità di un alleggerimento del Patto di stabilità interno è conosciuto da tutti e la

Stiamo parlando di migliaia di Comuni che non riescono più ad avere una boccata di ossigeno per andare avanti; stiamo parlando di dati - e sono dati ufficiali che nei primi otto mesi del 2009 sono saltati, in base a questa legge ingiusta del Patto di stabilità, 2.150 bandi pubblici proprio in un momento in cui la situazione economica richiederebbe iniezioni di sostegno e di rilancio all'economia delle piccole opere pubbliche e delle realtà municipali. municipali. Signor Presidente, signor Vice Ministro, immagino già la risposta che il vice ministro Vegas darà a questo emendamento, adducendo la necessità del rispetto di vincoli ed obblighi europei. Certo,

che lo sblocco dei residui del 4 per cento a favore dei residui passivi dei Comuni si è rivelato del tutto insufficiente e quindi è necessario che almeno in questo senso si incominci a alleggerire la morsa del Patto di stabilità. I Comuni hanno già dato. Il saldo dei Comuni è in attivo di un miliardo di euro. I Comuni I Comuni rappresentano soltanto il 2,7 per cento del debito pubblico complessivo delle amministrazioni locali. Credo quindi che la sensibilità di tutti i parlamentari, molti dei quali molti dei quali sono stati autorevoli sindaci nelle loro rispettive realtà territoriali e quindi conoscono la drammaticità che stanno vivendo attualmente le

*(PD)*. Signor Presidente, colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, quanti di voi nel corso di questi ultimi dieci anni si sono trovati di fronte un sindaco che lamentava il carattere stupido del Patto di stabilità interno? Dovendo esso essere organizzato attraverso una regola di tipo universale, che non distingue tra Comune e Comune,

uno strumento e una camicia di forza che impedisce loro non di assaltare la finanza pubblica e di metterla in pericolo ma, al contrario, di confermare il loro Comune in una scelta di stabilità e rigore finanziari, promuovendo però lo sviluppo della propria comunità. Quando discutiamo con questi sindaci - credo che capiti a me come a tutti voi Quando discutiamo con questi sindaci - credo che capiti a me come a tutti voi - diciamo loro: non potete pensare che il nostro Paese possa fare a meno di avere un Patto di stabilità interno, che collega la finanza dello Stato centrale a quella delle autonomie locali in modo tale che assieme possano rispettare i vincoli del Patto di stabilità esterno, quello che ci lega agli altri Paesi europei.

dalla sua modificabilità, sì, ma soltanto attraverso il concorso di tutte le parti che hanno concordato la sua definizione in passato,

signor Presidente, mi consenta l'espressione - i sindaci bravi escono di testa quando scoprono che due anni fa per rispettare il Patto di stabilità interno hanno fatto una cosa che, a causa del cambiamento delle regole, due anni dopo - credo di avere qui davanti uno di questi sindaci si è rivelato un comportamento irragionevole, assurdo e penalizzante per il Comune. Il sindaco dice: ma non potete trattarmi così! Sono il sindaco di un ente autonomo; se un anno mi dite che devo comportarmi in un certo modo per essere virtuoso, non potere trasformare la virtù del comportamento di quell'anno nel vizio tra due anni perché cambiate le regole. Sulla base di queste valutazioni - che come vedete anche in questo caso non hanno niente a che fare con le tecnicalità e le cose incomprensibili,

quando discutemmo in Commissione bilancio del disegno di legge Azzollini, proponemmo uno sforzo nella legge di contabilità per fissare alcune regole durature nel tempo, in maniera tale che quelle non cambino. Poi, gli obiettivi numerici del Patto di stabilità devono cambiare, perché la situazione economica e la realtà di finanza pubblica cambiano ogni anno ed è chiaro che ogni anno bisognerà avere un aggiustamento; ma le regole, non gli obiettivi quantitativi, del Patto di stabilità interno devono essere fissate una volta per tutte. Allora dicemmo: affrontiamo il tema della spesa in conto capitale e per quella parte, fissato l'obiettivo quantitativo alla dimensione nazionale nella legge di stabilità - attualmente nella legge finanziaria e prima ancora nella Decisione di finanza pubblica in termini di saldo complessivo

creato le condizioni politiche e amministrative necessarie per compiere questo investimento. Il Comune A ha nella sua Regione confinante un Comune B che dovrebbe fare l'investimento, ma che non rispetterebbe i vincoli del Patto di stabilità interno se lo facesse subito; allora il Comune B abbiamo scritto nella legge di contabilità - per regola data una volta per tutte può comprare il titolo d'indebitamento dal Comune A, il quale naturalmente riceverà indietro il titolo d'indebitamento quando negli anni futuri deciderà di fare il suo investimento. Attraverso questo meccanismo regolato a dimensione regionale - che, tra l'altro, è stato introdotto

di mettere in atto - che risultato otteniamo? Quello di rendere meno stupido il Patto di stabilità interno - mutuando l'espressione che usò Prodi a proposito del Patto di stabilità esterno - cioè consentire ogni anno

perché sappiamo quanto ci sia bisogno di investimenti nel sistema delle autonomie per la infrastrutturazione materiale e immateriale del nostro territorio. La norma che avevamo ipotizzato al Senato e approvato all'unanimità con il

modificare, ma sopprimerla completamente non è ragionevole: è un danno per il Paese perché in tal modo di nuovo il Patto di stabilità interno dei prossimi anni sarà caratterizzato da regole

Signor Presidente, il mio parere è contrario. Ci sarebbe naturalmente una discussione da fare, come abbiamo fatto per altri emendamenti. In questo caso, però, ritengo che sia più utile che sia il Governo a dare una risposta

Non poteva essere diversamente perché questa legge, innovando rispetto al passato, fa un bilancio che è leggibile attraverso tutta la pubblica amministrazione, non più solo al settore statale. Il comma 4, a mio sommesso avviso, non è modificabile. Diverso è il ripristino dei commi 6 e 7 i quali, in realtà, facevano un'operazione di iscrizione nella legge di contabilità di una regola che più opportunamente, in base alla legge n. 42 del 2009, dovrebbe essere oggetto del Patto di convergenza più che della legge di stabilità.

sia destinata ad essere modificata. Comunque, è meglio che questo tipo di regole vada a finire nel Patto di convergenza, cosa che deriverà dall'applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per questi motivi, mi permetto di invitare i presentatori a non insistere sulla votazione

rientro da un debito pubblico molto elevato, che altri Paesi europei hanno compiuto nel corso di questi anni, dimostra in modo ineccepibile che, quando si vuol fare fronte ad un debito pubblico molto elevato

programmare nel lungo e anche lunghissimo periodo come far fronte al debito e regolare la decisione annuale di spesa, naturalmente in rapporto all'entrata, cioè l'utilizzo del reddito annuale in rapporto a quel disegno di risanamento Queste esperienze ci hanno indotto, durante la discussione al Senato di questo provvedimento, a proporre che, nella definizione delle scelte fondamentali di finanza pubblica, che avvengono non nella legge finanziaria annuale - oggi legge di stabilità

programmatici non siano più espressi soltanto in termini di saldo. Saldo netto da finanziare, fabbisogno, indebitamento, sono tutti saldi, cioè rapporti di cassa, di competenza, come volete - ma pur sempre rapporti tra entrate e spese. È indispensabile, se si vuole far fronte e impostare addirittura un'azione di lungo periodo di risanamento, che gli obiettivi, che certo poi si definiscono anche attraverso il saldo, siano espressi partitamente, distintamente, in obiettivi di entrata e obiettivi di spesa. spesa. Questa decisione è cruciale, perché se l'obiettivo è espresso in termini di saldo può accadere, colleghi della maggioranza, quello che in particolare voi avete rimproverato ai Governi di centrosinistra, cioè che l'azione di risanamento venga condotta esclusivamente dal lato delle entrate, aumentando queste ultime e lasciando inalterato l'andamento delle uscite, cioè della spesa pubblica. La spesa corrente primaria nel corso degli ultimi otto anni, colleghi, è aumentata del 2,3 per cento all'anno, quale che fosse il Governo del momento. Questo ci dice

e che gli obiettivi siano vincolanti. Noi dicevamo a soli fini conoscitivi, non vincolanti per la definizione della legge di stabilità. Chiariamo nella Decisione di finanza pubblica qual è l'obiettivo di spesa globale, qual è l'obiettivo programmatico di spesa primaria e, di conseguenza, qual è l'obiettivo di pressione fiscale programmatico che ci diamo. La decisione della Camera è stata quella di abolire il riferimento alla necessità a fini conoscitivi di dare conto degli obiettivi distinti. Io, sinceramente, non capisco il perché. O meglio lo capisco, la ragione mi preoccupa sulla base di questa preoccupazione, ho ripresentato l'emendamento 10.6, che sarebbe, per la salute della Nazione, necessario approvare.

al comma 3, prevede che la legge di stabilità «non può contenere norme di delega» - e fin qui siamo all'ovvio - «o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio».

Il testo della Camera a questo punto si presenta in modo tale che, a mio giudizio, una interpretazione corretta del testo è che nella legge finanziaria non possono andare norme di carattere ordinamentale e organizzatorio che abbiano un impatto

l'intenzione che si voleva proporre, perché è del tutto evidente che nella legge finanziaria, signor Presidente, le norme ordinamentali che hanno un impatto

In questo caso però è possibile che l'interpretazione che darà il Governo come pacifica di questa norma possa essere sufficiente per dare l'idea che in realtà le norme che hanno un impatto sui saldi in legge di stabilità ci possono andare. Non sto parlando delle norme di sviluppo, ma delle norme ordinamentali con effetto sui saldi a partire dal primo anno di programmazione; è del tutto evidente, quindi, che la legge di stabilità deve avere la possibilità di contenere quelle norme. ecco perché ho presentato l'emendamento - che questa interpretazione benevola fosse solo mia e che, in realtà, restasse stabilito che la legge di stabilità non può fare ciò perché le norme ordinamentali con effetto sui saldi possono essere inserite solo nel collegato ordinamentale; potendosi presentare il collegato entro il 17 febbraio, faremmo uscire dalla sessione di bilancio le norme che hanno impatto sulla predisposizione del bilancio, il che, patentemente, è una soluzione priva di senso.

abbastanza obiettiva della norma mi porta a dire che la limitazione nel testo riguarderebbe esclusivamente le misure di carattere espansivo. Per questo motivo

quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio»: ciò vuol dire che queste norme non impattano sui saldi, quindi sono escluse, ad eccezione, però, di quelle che riguardano il Patto di stabilità interno. In questo caso possono essere anche previste delle norme di carattere ordinamentale o organizzatorio. A parte questo caso, la legge di stabilità regola semplicemente le grandezze,

*(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiarito il punto che il Governo ha il diritto di governare e padroneggiare la finanza pubblica il Parlamento ha il diritto e il dovere di controllare e chiarito che la certezza dei dati di finanza pubblica è un bene pubblico collettivo e, quindi, non riguarda maggioranza e minoranza nelle varie evoluzioni di una alternanza politica, il nodo centrale è se i dati di riferimento si debbano limitare ai saldi di finanza pubblica o debbano necessariamente rendere espliciti gli andamenti delle entrate e delle spese. spese. La legge n. 468 del 1978 fece, purtroppo, la scelta di limitare questo controllo ai saldi di finanza pubblica. ho già detto in precedenza, nonostante questo, quei saldi, nei trentuno anni passati, non sono stati tenuti sotto controllo, ed il risultato è il raddoppio del debito pubblico rispetto al PIL. Oltre a questo, in quegli stessi anni (vigente la legge n. 468) la spesa pubblica è aumentata di 7 punti di PIL e le entrate sono aumentate di 10 punti di prodotto interno lordo, cioè è cambiato il rapporto fondante del patto civile tra Stato e cittadino. Il peso dello Stato è aumentato di 10 punti; il peso dei liberi cittadini si è ridotto di 10 punti nell'ambito delle scelte quotidiane che ciascuno fa ogni giorno. Questo è il dato politico. Nel codice genetico del Popolo della Libertà, nel programma del Governo Berlusconi, il punto di fondo politico, promessa agli elettori per la quale abbiamo avuto un largo consenso, è quello di spostare questo confine: ridurre il peso dello Stato e ampliare la libertà di scelta e di decisione dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Questo è il nodo politico che il Popolo della Libertà e il Governo Berlusconi hanno posto al centro del proprio programma politico. È evidente che questo spostamento a favore della società, dei cittadini, in riduzione del peso dello Stato (che vuol dire Stato, Regioni, Province, Comuni e tutti gli altri enti della pubblica amministrazione) deve avvenire garantendo i saldi finanziari, cioè garantendo l'equilibrio finanziario; non può ridursi la pressione fiscale aumentando il deficit pubblico. Quindi, aritmetica vuole che per ridurre la pressione fiscale occorre ridurre il peso dello Stato, cioè la spesa corrente. Allora, la domanda che ci si pone in questa legge di riforma - che senza questo punto è legge di conferma della legge n. 468 e non di riforma aveva avuto nell'Aula del Senato una duplice risposta: da un lato quella di ottenere questa trasparenza e certezza dei conti pubblici espressi nei saldi, nelle entrate e nelle spese, attraverso l'unificazione dei Servizi bilancio di Camera e Senato e attraverso la Commissione bicamerale, non per il controllo, ma per la trasparenza dei criteri e dei metodi di determinazione dei dati della finanza pubblica. Questa era una strada, sulla scia, come è già stato detto, del *Congressional budget office*.

assegnare ad un'alta Autorità sulla finanza pubblica il compito di certificare tutti i bilanci delle pubblica amministrazione. Si tratta di una certificazione che giustamente chiediamo a qualunque impresa voglia quotarsi in borsa

che intermedia metà dell'economia nazionale non è certificato da nessuno ed è soggetto all'arbitrarietà di quei criteri di calcolo e agli andamenti tendenziali di cui abbiamo parlato in precedenza in quest'Aula.

contro il quale un'esigua minoranza che non accetta il risultato delle urne elettorali attacca in modo indegno, ora anche fisico, il nostro Presidente del Consiglio,

da parte dello Stato e di tutti gli enti della pubblica amministrazione, non semplicemente in astratto, ma nel concreto del netto in tasca che rimane a fine mese a ciascun cittadino italiano. Vi Vi chiedo questo. Lo strumento per razionalizzare la spesa pubblica è certamente l'avvicinamento della responsabilità delle entrate alla responsabilità della spesa. Si chiama federalismo fiscale. Questo è lo strumento che, nel tempo, dovrà produrre efficienza ed efficacia, in modo che ogni pubblico amministratore risponda con la propria faccia delle spese che fa e delle tasse che raccoglie. Ma se non poniamo questa pietra miliare, questa pietra d'angolo, come riusciremo a realizzare l'obiettivo del federalismo? Come arriveremo a definire quello strumento vitale per il futuro della Repubblica italiana in termini di democrazia partecipata, se nel frattempo confermiamo che la politica economica si limita ai saldi finanziari, non definisce i profili delle entrate e delle spese e non distingue fra spesa primaria e spesa per interessi? Ecco il senso della mia proposta, visto che la Camera ha modificato e stravolto questo punto, ossia il Servizio bilancio unificato e bicamerale sulla trasparenza. Perché non immaginare invece una Autorità indipendente che risponda al Parlamento, al Governo e al Paese? Prendo atto comunque che l'unanimità della Camera pesa e conta di più dell'unanimità del Senato, forse perché nell'unanimità della Camera qualche burocrazia autoreferente è riuscita a infilare con una microchirurgia distruttiva i propri interessi di conservazione di potere discriminatorio nella indicazione dei numeri. *(Applausi dal

proprio alle fondamenta di questa legge. Non credo che altri possano padroneggiare i conti pubblici che non siano l'Esecutivo, cioè il Governo, e il il Legislativo, ossia il Parlamento. Credo che i conti pubblici debbano essere affidati a queste due grandi istituzioni. Ne esiste una di controllo che è la Corte dei conti, la quale è l'unica ad avere carattere burocratico proprio perché svolge solo il controllo. Credo che non possiamo in alcun modo derogare dal principio dell'appartenenza dei conti pubblici alle espressioni, ai poteri democraticamente eletti.

si opponga all'elaborazione, alla classificazione e alla illustrazione dei conti pubblici in maniera distante dall'Esecutivo e dal Legislativo. Non credo che ciò sia possibile, nemmeno in via di principio. e delle finanze*. Il parere è ugualmente contrario, proprio per le considerazioni svolte dal senatore Azzollini. Quando si dice che l'Autorità ha il compito di verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario, oppure che l'Autorità fornisce una valutazione degli indicatori, vuol dire che questa sorta di tecnostruttura si sostituisce al Parlamento. Vale solo la pena di ricordare che i Parlamenti esistono perché nel 1215 Giovanni Senza Terra concesse la *Magna Charta* ed esistono per controllare le spese dei Governi. Se queste spese vengono controllare da una tecnostruttura mi domando quali siano gli effetti sulla democrazia. faccio solo presente che questo emendamento prevede una spesa di 100 milioni di euro, cifra che al vecchio conio sono 200 miliardi di lire, e mi sembra, se non ricordo male, che il famoso CBO americano

non si deve stupire della presentazione di questo emendamento e della proposta di introdurre nel nostro ordinamento la presenza di questa Autorità dei conti pubblici. Infatti, delle due l'una:

viene posta in capo al Parlamento (e io sono per tale soluzione, tant'è che avevamo adottato avevamo adottato e abbiamo riproposto in questa sede la scelta di dar vita alla struttura unica del Servizio del bilancio del Parlamento italiano),

perché nella forma di Governo neoparlamentare che abbiamo adottato dai primi anni Novanta in poi in Italia credo che la soluzione migliore sia

questa attività ha bisogno di strutture tecniche di elaborazione (che sono, in un caso, il CBO e in Italia per la nostra proposta potrebbe essere quella struttura unificata del Servizio del bilancio di cui abbiamo tante volte parlato). Quando si dice di no alle soluzioni più positive, più condivise e ragionevoli, naturalmente si spinge verso soluzioni che non sono condivise, magari come in questo caso della proposta dell'Autorità,

i decreti delegati attuativi della legge n. 42 del 2009 sul federalismo. Per questa ragione non parteciperò al voto su questo emendamento, perché la soluzione non mi convince, ma segnalo che essa, ove non

di un'autorità già esistente che regola i rapporti fra Governo e Parlamento oppure la costituzionalità delle leggi. Questa è una materia regolata dell'articolo 81 della Costituzione e l'unica autorità indipendente che esiste è la Corte costituzionale; tutte le altre autorità che entrano sullo stesso campo sono a mio giudizio pericolose. Per tale

Stiamo discutendo la legge di contabilità e finanza pubblica - ed abbiamo ascoltato in quest'Aula anche alcune lezioni per quanto riguarda la pubblica finanza anche per ridurre il peso dello Stato ed ampliare le libertà delle aziende e dei cittadini alla libera intrapresa. Questi sarebbero i princìpi delle economie e dei Governi cosiddetti liberali. Peccato, signor Presidente e colleghi, che tali princìpi spesso vengano calpestati. Come si concilia infatti la libertà d'impresa con il comma 79 dell'articolo 2 della finanziaria che per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge blocca tutte le azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali da parte dei fornitori? Mi riferisco a 18.000 aziende, spesso alla canna del gas per la crisi economica, che vantano crediti per 49 miliardi euro. Una norma europea recepita nella legge n. 23 del 2002 prevede i pagamenti entro 30 giorni;

lei ha richiamato poco fa Giovanni Senza Terra e - se non ricordo male - anche la Guerra dei trent'anni: non vorrei che questi emendamenti presentati portino ai pagamenti di 30 anni da parte della pubblica amministrazione; me lo consenta, perché voi parlate di liberalismo e poi eseguite norme contro il diritto liberale.

poco fa il vice ministro Vegas ha ricordato uno dei ruoli importanti del Parlamento che è quello del controllo dei conti pubblici. Allora, se uno dei punti prioritari della politica economica di questo Governo, così come è ribadito più volte nel Documento di programmazione economico‑finanziaria, è la stabilizzazione dei conti pubblici, non occorre una grande competenza in scienze economiche per comprendere che questo obiettivo di stabilizzazione può essere raggiunto attraverso due possibilità: l'aumento delle entrate o la diminuzione delle spese. Poiché l'aumento delle entrate nel nostro Paese è improponibile dato che abbiamo già una pressione fiscale devastante al 43 e poiché il problema della riduzione della spesa pubblica, che è un cavallo di battaglia che sta particolarmente a cuore al presidente Baldassarri poc'anzi ci ha ricordato l'ammontare del tetto complessivo della spesa pubblica che è sull'ordine degli 800 miliardi di euro), rivolgiamo un appello a una maggior attenzione dell'Aula su un altro aspetto che potrebbe consentire una stabilizzazione, sia pure a medio periodo, dei conti pubblici: questo aspetto è una vera lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Secondo dati, non nostri, ma del Ministero dell'economia, l'economia sommersa nel nostro Paese nell'anno precedente ha rappresentato il 18 per Stiamo parlando, per dare cifre e valori, di un gettito di oltre 100 miliardi di euro. euro. La Corte dei conti ha già più volte, in ripetute relazioni (l'ultima è quella del 2008), ribadito il fatto che la lotta all'evasione fiscale sta mostrando delle smagliature derivanti anche da recenti provvedimenti presi dal Parlamento, a partire da

pensa, noi vogliamo cogliere l'appello del vice ministro Vegas, che richiama il ruolo del Parlamento al controllo dei conti pubblici, chiedendo con l'emendamento

pubblica, con una relazione sia sui risultati effettivi della lotta all'evasione fiscale che sulle misure intraprese per migliorare l'efficacia e l'efficienza di questa lotta. Probabilmente si risponderà che la possibilità di avere da parte del Parlamento una relazione sulla lotta all'evasione è già un dato acquisito. In realtà non è così è bene che i colleghi richiamino la loro attenzione sul fatto che non è così. Infatti, la legge n. 296 del 2006, che ha consentito al ministro Padoa-Schioppa di riferire per la prima volta al Parlamento

dal ministro Tremonti in maniera piuttosto blanda: la relazione è stata presentata al Parlamento in maniera tardiva e forse c'è stata disattenzione e distrazione da parte nostra su un argomento particolarmente delicato proprio se si vuole raggiungere realmente questo obiettivo

infatti, l'articolo 17 riguarda le corrette modalità di copertura finanziaria delle leggi. Onorevoli colleghi, in ogni momento della nostra vita di Assemblea legislativa

o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

con introiti, cioè con aumenti di entrate, che si determinino una volta sola, perché tra la natura della copertura e la natura dell'onere c'è in quel caso assoluta incompatibilità. Con una decisione che io considero letteralmente incredibile - non so usare un altro aggettivo - la Camera dei deputati ha eliminato le parole «o non ricorrenti», con il risultato che, secondo la legge di contabilità, si può coprire correttamente un onere di parte corrente con entrate non ricorrenti. Questa si chiama dequalificazione gravissima del bilancio pubblico, non c'è un'altra definizione per questo tipo di scelta: se posso coprire con entrate *una tantum*, o che comunque si manifestano per un periodo limitato di tempo, oneri che si manifestano per sempre, naturalmente arrivo ad una dequalificazione del bilancio, perché nel primo anno l'onere sarà affrontato con risorse reali, ma nel secondo e nel terzo, quando le entrate non ci saranno più, l'onere permarrà: il risultato sarà un aumento del deficit e, di conseguenza, anche del volume globale del debito. In un Paese con un volume globale del debito come quello dell'Italia, questa è una decisione che non esito a definire irresponsabile: per questo motivo, ho presentato l'emendamento 17.2, che ripropone l'espressione «o non ricorrenti» tra le forme di copertura vietate.

trasparenza delle fasi di decisione nella sessione di bilancio, si tratta di un altro tema di enorme rilievo. Attraverso una prassi consolidata qui al Senato, che poi - che io sappia - si è estesa anche alla Camera, sia pure senza modificare di conseguenza né i Regolamenti né la legge di contabilità, in questa - abbiamo stabilito che l'obbligo di relazione tecnica per misure onerose (proposte emendative o disegni di legge) si estendesse da quello già previsto per il Governo nella legge di contabilità anche alle proposte avanzate dal relatore. E lei, signor come vanno le cose, lo sappiamo tutti: quando c'è una ragione di qualche imbarazzo politico per cui la proposta non può essere avanzata - per mille ragioni - dal Governo,

Che l'obbligo di relazione tecnica previsto per le proposte legislative onerose del solo Governo dovesse essere accompagnato dall'obbligo di relazione tecnica per le proposte del relatore:

nella quale l'obbligo di relazione tecnica non c'è per proposte che in realtà sono del Governo, ma che vengono avanzate dal relatore. Qui al Senato - e il presidente Azzollini, se vorrà, potrà darmene atto - siamo giunti addirittura a condividere

Questo forse lo otterremo chissà tra quanti anni, ma che almeno sugli emendamenti del relatore ci sia la relazione tecnica è una soluzione assolutamente ragionevole e utile per la qualità del nostro lavoro, nella sessione di bilancio in particolare. Propongo quindi l'emendamento che riafferma questo obbligo di presentazione della relazione tecnica anche nel caso della proposta del relatore. Infine, do per

ultimi trent'anni il debito è raddoppiato, le entrate sono aumentate di dieci punti di PIL e la spesa di sette punti, quindi la sua posizione precedentemente espressa è totalmente fuori luogo e non dimostrata da riscontri storici.

è il trucco attraverso il quale negli ultimi trent'anni si è aggirato l'articolo 81 della Costituzione. Nel lontano 1978, senatore Cabras (Presidente del Consiglio era un suo noto conterraneo), le forze sociali chiesero il raddoppio degli assegni familiari. L'onere in relazione tecnica era allora di 3.500 miliardi di lire perché il raddoppio era facile calcolarlo. La soluzione tecnica aggirante l'articolo 81 fu quella di procedere al raddoppio degli assegni familiari a partire dal 30 novembre, per due mesi nell'anno, quindi con 700 miliardi soltanto di entrate *una tantum* per quell'anno una spesa notoriamente pari a 3.500 miliardi. Questo esempio lastrica la strada del dissesto dei conti pubblici di questi ultimi trent'anni. Questo è proprio il trucco attraverso il quale non c'è trasparenza nella finanza pubblica, controllo da parte del Parlamento e assunzione di responsabilità da parte del Governo. Questa è l'essenza di questo piccolo emendamento che reintroduce, ancora una volta,

quanto riguarda gli oneri di parte corrente da coprire con entrate non ricorrenti, osservo solo che, certo, è un principio di grande rigore quello che avevamo espresso; pur tuttavia, la posizione della Camera non supera l'elemento fondamentale: se una spesa corrente è *una tantum* può essere coperta con un'entrata corrente *una tantum*; se è strutturale, non temporanea, allora anche l'entrata deve essere strutturale, non temporanea e sempre di parte corrente. In particolare, sul piano della competenza finanziaria la soluzione adottata dalla Camera è corretta. Quella adottata dal Senato era certamente più rigorosa, ma ma ciò non esclude la legittimità di quanto dalla Camera ci è pervenuto. Si tratta di un classico caso su cui si potrà discutere insieme in seguito, ma anche qui non c'è nessuna obiezione di principio al fatto che una spesa corrente

Per quel che riguarda, invece, la seconda questione, non c'è dubbio che una delle tecniche per tentare di evitare la relazione tecnica nel passato è stata quella di far di far sottoscrivere un emendamento dal relatore piuttosto che dal Governo, ma devo dire che più volte, nel caso in cui ci siamo resi conto di essere in presenza di emendamenti del relatore di una certa entità, abbiamo chiesto al Governo la presentazione della relazione tecnica. Questa non costituisce una prassi regolamentare, ma è stata una soluzione che, svariate volte, abbiamo adottato. Ma vi è di più. In questo testo, dell'articolo 17, viene espressamente previsto che i «Regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3». Dico sin d'ora che sarebbe opportuno prevedere nel Regolamento che gli emendamenti del relatore siano altresì corredati

nei Regolamenti parlamentari che si occuperanno di questo problema sia esplicitamente previsto che anche gli emendamenti del relatore siano corredati da relazione tecnica. Già che ci siamo, Presidente, siccome c'è un ulteriore tentativo

anche gli emendamenti di iniziativa parlamentare che rivelino una particolare complessità sotto il profilo finanziario siano accompagnati da relazione tecnica. Per questi motivi, il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti

alla relazione tecnica, sono perfettamente d'accordo con il presidente Azzollini: saranno i Regolamenti parlamentari a verificare, perché ci potrebbero essere emendamenti non presentati dal relatore, ma da un parlamentare destinati a passare e quindi a creare danni.

Collega Segretario, posso chiudere la votazione? Lei sta girando tutti i banchi o va in un posto ben preciso?

Colleghi, se vi accomodate questo controllo risulta più facile. Se lo complicate, non è che il controllo si interrompe: dura di più.

voglio segnalare a quest'Assemblea, alla sua attenzione in particolare e all'attenzione del Ministro competente la difficile situazioni in cui versa la società Yamaha Motor Italia. La Yamaha è *leader* nel settore della produzione di moto e di prodotti per il motociclismo ed è una delle aziende piccole, ma molto vivaci, ubicate nel territorio della provincia di Monza; la sede italiana si trova esattamente a Gerno di Lesmo.

Vorrei richiamare l'attenzione di tutta l'Aula e del Ministro competente sul fatto che in questo momento nell'azienda è in atto una vera e propria serrata, per cui gli operai, ancorché ancorché soggetti al licenziamento (ma la procedura non è ancora ultimata), non possono entrare in azienda. Alcuni di essi hanno occupato lo spazio del tetto

a sottoporre l'azienda ad un procedimento diverso; quindi, gli stessi imprenditori sono del parere che valga la pena accertare se sussistono le condizioni per potere ricorrere all'utilizzo della cassa integrazione. Ovviamente il sindacato ha molto sostenuto questa posizione, ma la proprietà della Yamaha non intende recedere. È chiaro che siamo in presenza di una difficoltà - se vogliamo - di carattere legislativo,

Pertanto, chiedo, da un lato, una risposta immediata all'interrogazione da me presentata, unitamente alla senatrice Baio, in data 26 novembre.

di fare quanto possibile per intervenire su queste aziende al fine di evitare che la produzione cessi così drasticamente. Soprattutto, gli operai non sanno che cosa fare perché la cessazione dell'attività

finora ha cercato, pur con tutte le difficoltà, di salvaguardare posti e di non creare problemi eccessivi al Governo.

Signor Presidente, intervengo in merito al preannunciato giro di vite su Internet a seguito del gesto compiuto a Milano contro il Presidente del Consiglio. questo perché le agenzie ci informano che il ministro Maroni ha annunciato che un decreto-legge apposito dovrebbe essere discusso nel prossimo Consiglio dei ministri. Questo è un Paese che si fonda *in primis* sulla non certezza del diritto, e quindi qualsiasi tipo di norma deve avere sempre a che fare con il fatto che è talmente violatrice dei nostri principi costituzionali che applicarla è un disastro. Ma questo è anche l'unico Paese in Europa che, in primo luogo, ha criminalizzato una tecnologia, ossia lo scambio dei dati con il cosiddetto *peer-to-peer*; in secondo luogo, con il decreto Pisanu, ha imposto tutta una serie di vessazioni non soltanto a chi

con tutti i Governi, devo dire - negli ultimi dieci anni in relazione alle manifestazioni sportive, che oggi il ministro Maroni dice dovrebbero essere trasportate al dominio virtuale di Internet. In questi giorni abbiamo incardinato in 1a Commissione una revisione di alcune di dette norme che regolamentano l'accesso alle manifestazioni sportive, perché in effetti sono inapplicabili, oltre che incostituzionali. onde evitare di ritrovarci fra due mesi a dover approvare - come abbiamo già fatto - un emendamento del collega D'Alia per poi farlo cancellare dalla Camera dei deputati dagli stessi che lo avevano suggerito alla maggioranza (tramite però un membro non della maggioranza), sarebbe il caso di bloccare ogni provvedimento che vada a creare uno Stato di polizia sul modello cinese o iraniano in Internet, aprire un dibattito in 1a e 2a Commissione, magari coinvolgendo anche le altre (non saprei però quale Commissione è competente su Internet, perché la materia mette insieme molti aspetti), coinvolgere chi la rete la conosce e non esclusivamente dal punto di vista legale ma da quello della vera legge della rete, ossia i codici, ed eventualmente, nelle prossime settimane o alla ripresa dell'anno prossimo, finalmente svolgere un dibattito parlamentare nel merito e nel metodo della presunta

Paese che eccelle nell'ingegneria elettronica, in particolare nel campo di Internet e di tutto ciò che attiene ai *software* che questo possono anche regolamentare e far crescere. Se non ci dovessero essere

di oggi: stanotte un altro matto voleva andare nella camera del presidente Berlusconi ed è stato fermato dalle forze di polizia. Credo che questo matto

«La Sapienza», che viene a costare all'Erario, quindi a noi, il 20 per cento in più ed elimina 12 piccole aziende che lavorano già all'interno del Policlinico. Tutto ciò è stato progettato per dare la possibilità ad una grande cooperativa